e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. **Preannunzio di votazioni

2, che recita come segue: «Revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata

ha pensato di tener conto solo di alcuni nel dibattito e non di altri

Presidente, i dibattiti parlamentari servono ovviamente anche per ascoltarsi e per ascoltare le ragioni reciproche; non è che si deve necessariamente trovare una mediazione, ma questo serve per ascoltare le diverse osservazioni. Mi pare che la proposta della relatrice si faccia positivamente carico di questo dibattito, senza alcun cedimento rispetto alla proposta del Governo, che parlava di eliminazione graduale.

della presenza degli animali nei circhi. Quindi mi pare che, mettendo insieme questi due principi (l'estensione allo spettacolo viaggiante e il graduale superamento), si possa avere una norma ragionevole. Non so

di poter avere almeno un'ora di tempo e di sospendere la seduta, perché, come giustamente osservava il senatore Giovanardi, se dobbiamo stare qui e intervenire sugli altri emendamenti, non possiamo certo lavorare sui subemendamenti riferiti

teatro Eliseo perché, secondo la situazione che mi è stata rappresentata (ma non so se sia vera o no), ci sarebbe stato un impegno formale del Governo a finanziare il teatro Eliseo con 4 milioni di euro, che mi dicono sarebbero stati stanziati nella finanziaria, quindi sarebbe un dato certo. 2 di questi 4 milioni, giusto o sbagliato che sia, sono stati dirottati su spettacoli da tenere da parte delle Regioni nelle zone terremotate, quindi coloro che avevano l'aspettativa di ottenere questa somma se la sono trovata improvvisamente decurtata.

dei fondi stanziati per i diciottenni e per la cultura che non sono stati ritirati e che quindi sono a disposizione. Queste sono le ragioni per cui ho presentato un emendamento sul teatro Eliseo. Eliseo. Se è vero che nella finanziaria una somma era stata stanziata; se è vero che è stato fatto questo affidamento; se è vero che sono stati fatti investimenti per 4 milioni di euro; se è vero che 2 milioni di euro sono stati sottratti e indirizzati da un'altra parte, mi sembrerebbe giusto ripristinarli.

che specificava che agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge

i bambini, magari nati in famiglie più disagiate e quindi anche con meno possibilità di iscriverli a questi corsi e mi si invita a chiedere al Governo di valutare l'opportunità? Ma quale opportunità? L'opportunità è già stata valutata, è una cosa da fare e non c'è da "valutare se farla":

tenevo a questo ordine del giorno, chiedo alla presentatrice di fare una riflessione ulteriore

un impegno a fronte della valutazione dei limiti della finanza pubblica con i quali il Governo in futuro si dovrà confrontare. Il Governo, quindi, è disposto ad impegnarsi ad acquisire questa sollecitazione e, compatibilmente con le altre emergenze che si presenteranno,

Presidente, non vorrei commettere uno sgarbo istituzionale nei confronti della relatrice, che si dimostra così aperta al dialogo e così ben disposta. So bene che tiene molto a questo tema,

per ottenere queste risorse. Pertanto propongo alla relatrice un'altra formula e vediamo se così riusciamo a trovare la quadra.

è tutta incentrata sull'emendamento del Governo e sui subemendamenti, i quali - che

verrà eliminata anche la possibilità di utilizzare o fare spettacolo con i cavalli e con i cani. Poi, naturalmente, ci sarà il problema degli animali selvatici, ma se concentriamo su quel subemendamento del Governo e sugli altri subemendamenti, almeno facciamo capire ai lavoratori dei circhi e agli italiani che cosa sta facendo

al testo che era arrivato in Aula e che tra l'altro era stato presentato dal Governo. È evidente a tutti che

potuto essere accettata solo nel caso in cui ci fosse stata chiaramente l'indicazione di un termine temporale, e non solo con l'aggiunta degli spettacoli viaggianti, che fa riferimento anche a questo mio emendamento. Questo termine temporale

anche della ricollocazione dei lavoratori, facendoci carico di un processo di riconversione; così come abbiamo presentato, a mia prima firma, un emendamento che

ripristinare il termine «eliminazione», ma indica anche una modalità premiale per i circhi e le attività che avviano la riconversione dando una premialità nell'accesso

perché quando diciamo che bisogna avviare rapidamente questo processo con una riconversione e con dei sostegni, lo facciamo anche perché tutti noi siamo coscienti della crisi profonda sta attraversando questo settore e pertanto, evidentemente, lo facciamo anche per il bene e il futuro non solo di quest'attività, ma anche di coloro che ci lavorano. Ci siamo invece trovati di fronte a una serie di distinzioni (cavalli, animali selvatici) e di discussioni che francamente sono soltanto segnate dal fatto che non si vuol avviare questo processo; in questo senso dispiace molto, moltissimo che il Ministro e la relatrice abbiano di fatto

Quale finalità hanno le corse dei cavalli se non il divertimento? Volete della socializzazione? Hanno una qualche funzione che non sia quella storica di una collaborazione uomo-animale per necessità? Secondo il ragionamento della collega, tutto questo dovrebbe essere eliminato. Non si possono usare i cavalli per il polo, non si possono usare i cavalli per l'ippica non si possono usare i cavalli per l'ippica o per il *dressage*, perché vengono addestrati per attività ludiche e la gente va a vedere le corse dei cavalli perché si diverte. Ma vi rendete conto di dove stiamo arrivando?

dell'utilizzo degli animali selvatici. Ma qui, signori, stiamo arrivando a teorizzare, ancora una volta, l'eliminazione di un rapporto di collaborazione fra l'uomo e l'animale, sostenendo, in alcuni emendamenti, che l'uomo può mettere a rischio la sua vita e può fare il trapezista, trapezista, può fare esercizi continui, ore ed ore al giorno, per guadagnarsi da vivere nel circo, ma l'animale no.

la ragionevolezza di emendamenti che semplicemente consentono al circo equestre - che tale si chiama - di continuare nella vocazione per cui è nato. Dobbiamo, quindi, consentire di fare gli spettacoli con i cavalli e con i cani, con quegli animali che collaborano con gli uomini e con le donne dappertutto, nello sport, nella cultura, nella necessità e nella disgrazia. Signor Presidente, ho sottoscritto alcuni subemendamenti del collega Giovanardi dopo un'attenta riflessione. Mi sono reso conto, infatti, che si è scivolati verso una forma di contrapposizione estrema, oserei dire integralista, su cui, invece, il buonsenso deve fare la differenza. Di conseguenza, invito l'Assemblea a riservare attenzione e ad entrare nel merito di questa deriva,

L'evoluzione che può di fatto determinarsi - qualcuno ha parlato del Palio di Siena, io parlo della Quintana, qualcun altro può parlare di tante altre cose - può riservare conseguenze critiche per il futuro non solo del Governo, ma anche del Parlamento. Dunque, attenzione, approfondimento e bando a queste forme di integralismo estremista, che sta emergendo

chiedo di poter sottoscrivere questo emendamento. Credo che siamo davanti alla necessità di prendere delle posizioni chiare rispetto a un tema che ha sollevato un grande dibattito

Continuare però con formule di mediazione, di trapasso e di superamento, credo sia veramente l'ennesimo segno della nostra incapacità

facciamolo entro una data e nell'emendamento propongo «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge». Nel frattempo avremo l'opportunità di valutare, dai casi più gravi

sono amareggiata anche per l'aridità di certe argomentazioni che sono state fatte, che dimostrano, come al solito, la mancanza di sensibilità in quest'Assemblea.

Questa era la direzione principale cui si mirava con questo testo e con quella frase, cioè la graduale eliminazione degli animali nei circhi. Quando parliamo di eliminazione degli animali nei circhi, pensiamo all'orso con il tutù che deve andare in bicicletta o all'elefante che deve stare su una zampa

Quelli di oggi saranno altri tipi di orrori, ma ogni volta che si sfrutta e si maltratta chi è più debole è sempre un orrore. un orrore. Concludo ricordando che più della metà dei Paesi europei oggi vieta l'utilizzo degli animali

ma siamo sempre allo stesso punto. La verità è che questo è un Paese vecchio, con una mentalità vecchia, che questo Parlamento rappresenta perfettamente. È un Paese conservatore, cui alcuni si dichiarano progressisti e non conservatori, e poi, ogni volta che c'è da fare un cambiamento, il coraggio viene sempre a mancare. Io invece voglio sperare lottando - per quel che valgo, cioè molto poco, quasi niente - per un Paese più aperto, che faccia dei cambiamenti in positivo, soprattutto per quel che riguarda certi principi di civiltà. Io penso che sia meglio valere poco, quasi niente, ma è meglio valere uno che valere

perché non mi è chiaro come si possa accettare un ordine del giorno che contiene esattamente le stesse affermazioni dell'emendamento della relatrice,

su come legiferare al meglio. Allora come si può mantenere un emendamento della relatrice con identico contenuto

sembra un controsenso. Siamo in grado di definire normativamente e con il linguaggio? Questo è il lavoro pesante che facevano anche i nostri padri Costituenti, cioè quello di discutere su un termine, ma poi trovavano la quadra. Qui invece si dribbla da una parte e dall'altra e non mi sembra che stiamo raggiungendo la definizione di un disegno di legge delega, che contiene questo e tanto

questa manipolazione semantica servisse per rasserenare il clima nell'opinione pubblica che ormai ci chiede di compiere questo passo. Quindi li rassereniamo in previsione delle prossime elezioni politiche e poi si vedrà, perché tanto «graduale superamento» non significa alcunché.

a quello che può pensare il ministro Franceschini, l'opinione pubblica italiana non è così ignorante da non capire che la gradualità non significa alcunché; se quindi spera di vendere questa fumata (di gradualità e superamento) a quello che lui spera sia il suo futuro

La colpa può essere del padrone, ma se un cane ha un dente cariato qualsiasi medico vi spiegherà che può essere educato finché volete, ma se è in una situazione di dolore, se qualcuno gli si avvicina, come un bambino, lo sbrana perché è un animale e non è in grado di connettere quando è in certe situazioni. Ma, ripeto,

che interessa una minoranza, anche culturale, avrebbe la maggioranza del popolo italiano contro, perché la sensibilità è farsi gli affari propri ed eliminare qualsiasi cosa che non piaccia. Ma in una società liberale non funziona così: così: chi non vuole andare a teatro non ci va, e credo sia giusto che lo Stato spenda dei soldi per mantenere una nota tradizione lirica, sinfonica e musicale, anche se da sola non si sostiene.

nel prevedere il graduale superamento dell'utilizzo di alcune specie di animali, mi sembra che lasci ampio margine al Governo nell'esercizio della delega per individuare, su solide basi scientifiche, quali specie sono incompatibili con l'attività circense e quale attività, invece, non reca alcun danno al benessere degli animali. Annuncio, quindi, il mio voto favorevole.

più. Lo stesso ragionamento, se me lo permettete, posso fare per il circo. Fra le altre cose, Pavarotti andava a cavallo e organizzava a Modena riunioni ippiche. Abbiamo anche ironizzato sul fatto che

un'eccezione per animali come cani e cavalli, abitualmente utilizzati in attività di spettacolo, sportive e di collaborazione con l'uomo. Come vedete, si fa una discriminazione odiosa

al guinzaglio? Non si può far fare a un cavallo un giro di pista? Stiamo scrivendo una cosa del genere? Diciamo almeno che questi animali, che abitano nelle nostre case e sono i nostri compagni, e sono così diffusi, possono continuare a lavorare anche nel circo, come lavorano in altri mille settori.

cari signori delle associazioni animaliste, che è ancora in vigore la vergognosa legge che permette alle associazioni animaliste di denunciare, anche penalmente, gli allevatori, i produttori e i circhi.

un *dossier* dell'Ente nazionale circhi, che stanno distribuendo, sulla montagna di menzogne (una valanga di bugie) raccontate da alcune associazioni. Lo vogliamo approfondire? Lo vogliamo leggere?

Votiamo questa norma, che secondo me fa anche un favore al Governo e alla maggioranza, perché in qualche modo salva la legge.

e che ha come protagonisti principalmente i cavalli, i cavalli dei Carabinieri, del reggimento dei Carabinieri a cavallo. Se non facciamo i conti

genere la sensibilità di molti di noi sia ai livelli più avanzati. Io rispetto gli animali, anzi li mantengo e non ne faccio un uso speculativo di alcun tipo, né di affezione e neanche economico. fanno parte del contesto naturale del nostro pianeta e come tali devono essere rispettati, come tutti gli altri esseri viventi, compresi le piante e i minerali (se vogliamo rispettare il nostro mondo, dobbiamo tener conto anche di questo). Ma io credo che ci debba essere una razionalità di comportamenti e di valutazioni per evitare contraddizioni enormi. La manifestazione della festa anniversaria dell'Arma dei Carabinieri è uno spettacolo

e la scienza ci può dare una grande mano, checché ne dicano i mangiati e vomitati di queste giornate

relativamente a spettacoli che non cagionino sofferenza agli animali e nello stesso tempo, nel momento in cui parte il

in relazione alla tipologia di utilizzo degli animali; identificare, parimenti, i criteri idonei ad identificare le tipologie di animali che possono essere più celermente dismessi dall'utilizzo in attività circensi e spettacoli viaggianti;

«il loro inserimento in specifiche aree e in strutture atte alla loro riabilitazione, ivi comprese, compatibilmente con le specifiche esigenze, le aree protette identificate nell'elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 6 dicembre 1994, n. 394, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il coinvolgimento del personale

Presidente, invito la relatrice e anche la senatrice Fucksia a rendersi conto di cosa significhi

si gestiscono il sistema delle aree protette e la biodiversità, la quale è molto delicata nel nostro Paese. Noi non siamo nella foresta amazzonica o in Africa.

natura linguistica: «revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante»,

intervengo per motivare il mio voto contrario su questo emendamento che in qualche modo imbroglia tutti: attraverso un artifizio letterale, cancella «eliminare», «eliminare», che si capiva cosa voleva dire, e usa il termine hegeliano «superare» - tesi, antitesi e sintesi - che non si capisce assolutamente cosa voglia dire, se non - come mi hanno riferito autorevoli giuristi del Consiglio di Stato - che è un modo diverso per dire «eliminare».

per trovare un compromesso e far passare la legge, facciamo una roba che non ha senso. Inoltre, si ribadisce il concetto filosofico ideologico di fondo di una visione della negazione assoluta del rapporto di lavoro dell'uomo con l'animale, in relazione anche a situazioni che riguardano

sorte toccherà anche al carosello dell'Arma dei carabinieri e a tutto quello che ha a che fare con il cosiddetto benessere animale che, però, ci si rifiuta di

Perché si esibiscono in pubblico? Ma anche quelli si esibiscono in pubblico quando vengono fotografati per propagandare la cultura animalista. E allora che facciamo? Facciamo le proibizioni selettive?

qui - il fatto che si teneva conto di una nuova sensibilità dell'opinione pubblica e della crisi del settore, cercando anche di avviare un processo di riconversione nel rispetto della dignità degli animali. Qui si sono dette delle cose ridicole. Si sono confusi i Carabinieri con le attività circensi; si sono fatte confusioni incredibili; si è arrivati al punto di accettare ordini del giorno per cui si possono mettere - ad esempio - leoni e coccodrilli all'interno del sistema delle aree del nostro Paese. Ciò è a dimostrazione, al di là dell'invocazione scientifica di qualcuno, che forse non ci si rende proprio conto. Qui non stavamo parlando di

volontà di arrivare effettivamente a una riconversione; si arriverà a distinguere tra animale e animale e probabilmente tutto questo finirà in niente. Questo

Allo stesso tempo, non pensiate che state facendo un favore al circo. Con questo atteggiamento non avrete certamente il merito di portare il circo fuori dalla crisi, perché state impedendo nei fatti e decelerando fortemente qualsiasi ipotesi

questo processo, ma non ne avete voluto tenere conto e siamo ridotti a fare una discussione legata a delle piccole pressioni, a piccole cose. Non vi rendete conto - lo ha detto benissimo anche la senatrice Repetti - che 15 Paesi in Europa hanno fatto questo percorso. Il Cirque du Soleil è

A causa di una serie di scioperi indetti da alcune sigle sindacali facenti capo ai Cobas, da circa dieci giorni sono in corso picchettaggi davanti agli *hub* della SDA, una delle più importanti aziende di logistica e spedizione italiane, con particolare riferimento agli *hub* di Bologna, Piacenza e Milano. Questi scioperi - la cui ragione rimane misteriosa rimane misteriosa (sembrerebbe legata ad uno scontro interno tra queste sigle per il controllo della gestione delle tessere sindacali all'interno dei lavoratori delle cooperative), stanno producendo un gravissimo danno ad un'azienda che è partecipata in maniera totale dalle Poste italiane. Siamo arrivati a 150.000 spedizioni ferme e 500 spedizioni non prese in carico. Ricordo che SDA lavora per moltissime e importanti aziende italiane e consegna i pacchi per Amazon. quindi rischiando un danno gravissimo, e soprattutto occupazionale in questo Paese, nel più totale silenzio. Purtroppo a cominciare da quello che sta avvenendo a Milano, dove stanotte c'è stato un blocco molto duro da parte di un gruppo di lavoratori, non c'è un intervento da parte dei prefetti delle città coinvolte. Rivolgo quindi un appello al Governo, al ministro Minniti in particolare,

Presidente, Honeywell di Atessa, in provincia di Chieti, è uno stabilimento sito nella zona industriale della Val di Sangro. Produce turbine per motori diesel e impiega circa 400 lavoratori. In tale stabilimento i lavoratori sono in sciopero a tempo indeterminato, utilizzando la loro ultima e disperata risorsa prima della chiusura della fabbrica. L'intenzione del gruppo che gestisce la Honeywell di Atessa è infatti quella di delocalizzare la produzione in Slovacchia, privilegiando un analogo stabilimento che si trova in Francia. Tutto questo avviene nonostante il fatto che la Honeywell di Atessa sia considerata un'eccellenza per qualità e professionalità, nonché un fornitore di importanza strategica per altre fabbriche dell'*automotive* presenti in Val di Sangro Quello che indigna di più è che i vertici della Honeywell, proprio per giustificare una decisione incomprensibile, parlano di motivi di sicurezza, con riferimento ai terremoti che negli ultimi anni hanno afflitto l'Abruzzo. A questo punto, dovremmo chiudere baracca e burattini, visto che l'Italia è quasi interamente un territorio sismico. Sentire scuse del genere mi fa male come abruzzese ed essere umano.

Purtroppo, parlando con i lavoratori della Honeywell proprio stamattina, ho appreso che il loro incontro al Ministero dello sviluppo economico è stato del tutto inutile, senza la presenza di dirigenti Honeywell di primo piano e senza concludere nulla di concreto.

sottolineo alla Presidenza l'urgenza di anticipare un nuovo e più risolutivo incontro fra Governo, dirigenti della multinazionale e rappresentanti dei lavoratori. Non si può chiedere a lavoratori già esasperati di aspettare ancora qualche settimana. Bisogna chiudere la questione subito e in modo efficace. Nei prossimi giorni sarò di persona al presidio dei lavoratori in sciopero ad Atessa. Bisogna parlarne il più possibile e nei titoli di giornale devono esserci anche e soprattutto queste storie vere e non solo i trionfanti dati teorici su PIL e occupazione. È una follia rinunciare a una fabbrica che funziona bene, abbandonando centinaia di lavoratori e le loro famiglie. *(Applausi del